Comunico che a nome del prescritto numero di senatori è pervenuta la richiesta di inserimento urgente nel calendario dei lavori dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 55, comma 7, del Regolamento, della discussione della mozione n. 813, e altre eventualmente abbinabili, concernente la responsabilità gestionale degli amministratori delle banche fallite. La votazione di questa richiesta avrà luogo al termine della seduta.

vorrei sommessamente far presente che la relatrice nel primo pomeriggio ha presentato

su cui il rappresentante del Governo ha espresso un orientamento favorevole, ma la Commissione bilancio ha chiesto la relazione tecnica per poter essere certa. siamo costretti a chiedere un accantonamento fintantoché non verrà resa la relazione tecnica, altrimenti il nostro parere resterà contrario.

il discorso è abbastanza irrilevante, perché se si fa la vaccinazione a dei ragazzi giovani, si presuppone che essi non siano immuni. Diverso è il discorso per gli adulti. si venga a fare il discorso della trasmigrazione degli anticorpi dalla madre al bambino, perché quell'immunità trasferita dura poco tempo e non a vita. Detto ciò, dobbiamo tener conto del fatto che

fare anche una formulazione monovalente.

e ovviamente i colleghi hanno ragione nel voler sapere da dove vengono questi soldi e se sono effettivamente disponibili. Qui c'è però un vizio di forma e di fondo nella relazione illustrata dalla relatrice, nel senso che che mi pare di non aver ascoltato quanto in questo momento apprendo - anche se per la verità l'ho appresso dalla stampa nei giorni scorsi - ovverosia che il Codacons ha finalmente ottenuto dall'Aifa i dati sulle reazioni avverse ai vaccini negli ultimi tre anni.

perché qui non stiamo combattendo la poliomelite come ai tempi eroici degli anni

da *deficit* di neurosviluppo. Malattie che sono specificamente collegate alla presenza di alluminio. alluminio. Se in quest'Aula non si ha la percezione che questo non è il gioco tra coloro i quali credono nella scienza e nei vaccini e i trogloditi, gli antiscientisti,

Senatore D'Anna, la richiamo all'ordine.

la cortesia di garantire il rispetto degli oratori. Il Ministro è presente perché ha una funzione di recepimento delle nostre istanze e non per produrre un effetto termico.

fanno parte della relazione che hanno tenuto sui vaccini o non ne fanno parte; omesso di informare il Parlamento su questi dati, avendo ricevuto, sia l'Aifa che la signora Ministra, una denuncia da parte del Codacons per omissione di rivelazione di questi dati. Sono 21.658 casi di reazioni avverse, di cui 454 gravi, in tre anni. Non stiamo parlando della pantomima di uno su un milione.

Abbiamo lavorato la scorsa settimana, nonostante tutto questo, accantonando una serie di emendamenti importantissimi, e ci ritroviamo oggi, all'apertura dei nostri lavori, con un punto

possiamo però utilizzare il tempo a disposizione per andare avanti su altri argomenti che non hanno alcuna connessione con tutto ciò che è stato accantonato.

Presidente, rispetto la sua decisione e, qualora fosse l'unica percorribile, andremo a verificare gli altri emendamenti.

Signor Presidente, mi dissocio dai toni e dai proclami su quelli che interverranno dopo. In coscienza, l'intervento della collega Taverna ha una sua razionalità:

la sua decisione, ma se ci viene chiesto un parere, visto che non lo abbiamo espresso, in coscienza devo dire che quanti chiedono una sospensione hanno un'oggettiva ragione e questo evidentemente indipendentemente dall'opinione completamente diversa che abbiamo sulla materia. [DE

decisione deriva dall'esame dell'articolo 2 che, trattando di iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni, non ha nessuna connessione

procedura. Tanto perché sia chiaro, i tempi a disposizione dei vari Gruppi sono già esauriti.

Signor Presidente, per la regolarità dei nostri lavori, vorrei dire che mi sembra che su questo ordine del giorno ci fosse stata una richiesta di votazione per parti separate

vaccinale. Questo innalzamento lo vedo anche in relazione alla necessità, visto questo carico di vaccinazioni obbligatorie, di una relazione più

Scilipoti, la richiamo all'ordine. Avete abbondantemente utilizzato il tempo

Quindi, prima di votare l'articolo 2, forse va verificato che il coordinamento sia giusto o errato, sennò poi rifacciamo la stessa cosa che abbiamo fatto dieci giorni fa in Aula, quando abbiamo espunto una parte del coordinamento e l'abbiamo dovuta trasformare in emendamento.

a mio parere rientra nella proposta di coordinamento, quindi non ci sono motivi ostativi a proseguire.

ordine del giorno.

Grazie,

Quindi le Regioni a Statuto speciale avrebbero un altro trattamento? Questo si vuol dire?

sarà lei a decidere se la volontà dell'Assemblea prevalga sul Regolamento, dovendosi rispettare la finalità che l'Assemblea intende perseguire, oppure se restringere il tutto dentro il perimetro, che nella fattispecie diventerebbe asfittico,

far prevalere la logica dell'informazione, della formazione e della sensibilizzazione sulla prevalente volontà di un'obbligatorietà che è stata introdotta nel provvedimento. L'emendamento 2.2 va proprio in questa direzione. Durante il lavoro in Commissione mi è stato chiesto di

seguenti «da svolgersi anche con la collaborazione». Ho ritenuto addirittura migliorativa la richiesta che mi è stata fatta dalla relatrice e dal Governo e, quindi, ho

Presidente, c'è un notevole livello di confusione intorno a questo elemento. Vediamo di fare un po' di chiarezza. Nel suo

quando ha messo in votazione questo emendamento, ha detto: «parere contrario». In questo modo, secondo una prassi assolutamente comprensibile, ha dato un'indicazione errata all'Assemblea. Ciò, dal mio personale punto di vista, inficia il voto che c'è già stato.

è stato bocciato dall'Assemblea. È chiarissimo e non c'è più niente da discutere.

Presidente: quell'emendamento è stato bocciato. La relatrice, la Commissione e il Governo devono trovare altre soluzioni, ma non si può tornare indietro, perché se torna indietro, signor Presidente, ciò significa che possiamo tornare indietro su tutti gli emendamenti che bocciamo.

aderito a una interpretazione magari legittima, ma certamente restrittiva, della portata regolamentare, con riferimento a un voto già espresso in esito a un parere del relatore. Mi riferisco al codice antimafia, votato la settimana scorsa. Ricorderà, signor Presidente, che, per un

causato da un parere espresso dal relatore e per un voto espresso, non si può tornare indietro, perché altrimenti del Regolamento del Senato, che - come lei sa - ci stiamo facendo parte diligente… ho appena detto che non torniamo indietro.

un tema al quale teniamo molto, perché si chiede al Ministero della salute di promuovere un'adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni. Perché l'ho ritirato? L'ho fatto perché, pur avendolo a lungo discusso in Commissione, su di esso era stato espresso parere contrario da parte sia della relatrice che del Governo. Quindi, nel tentativo di concentrare la discussione su alcune questioni che ritenevo fossero fondamentali, proposte che mi sembrava non avessero possibilità di essere accolte. Dopo di che la relatrice oggi ha detto - e il Governo lo ha confermato - che il parere è favorevole.

L'emendamento nasce con l'intento di specificare, laddove si dice che ai consultori familiari è affidato il compito di diffondere le informazioni relative alle disposizioni di cui al presente articolo,

ribadisce semplicemente che nei consultori si devono continuare a fare le vaccinazioni, piuttosto che farle fare in farmacia.

su questo argomento. Le cose sono andate come segue: la volta scorsa non abbiamo avuto modo di discutere questi emendamenti e, quindi, non eravamo a conoscenza dei vari ritiri. Il fascicolo è stato consegnato prima dell'inizio dei lavori,

prima c'è un ritiro e viene scritto sul fascicolo che l'emendamento è ritirato; viene negata alla senatrice Taverna la possibilità di farlo proprio e adesso lei dà la facoltà - la senatrice Dirindin non me ne voglia

la relatrice può presentare un emendamento a sua firma e tutti i Gruppi si impegnano a non chiedere tempi per subemendare. Se c'è l'impegno dei Gruppi a non subemendare, presento l'emendamento come emendamento della relatrice.

finestra"). L'emendamento serve a promuovere un'adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale. Mi pare che amplia molto

che nei consultori italiani, laddove c'è il decreto di autorizzazione e funzionamento ai sensi di legge - il che non è vero nell'80 per cento dei casi, e ne prenda nota chi deve farlo - non

Presidente, a beneficio del Resoconto stenografico, credo sia utile ricordare che, differentemente da quanto accade generalmente, i termini di scadenza per la presentazione degli emendamenti coincidevano sia per la Commissione che per l'Assemblea. Ed è questo il motivo per il quale noi troviamo all'esame dell'Assemblea anche emendamenti il cui testo è già stato superato durante i lavori in Commissione. Questo serve anche a far comprendere i testi riformulati che convivono con i testi originari, e non perché i proponenti abbiano inteso proporli all'Assemblea dopo il parere favorevole raggiunto in Commissione, ma perché i termini di scadenza previsti per la presentazione di emendamenti per questo, che è un decreto-legge, coincidevano. Accolgo l'invito di

Qui si tratta di indicazioni cogenti rispetto a dei comportamenti che sono conseguenti a delle scelte legislative e un ordine del giorno può essere proposto come intento. A parte il fatto che non riesco a capire

c'è scritto che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e tutoriale devono sottoscrivere apposito modulo. Non c'è solo quello che ha detto la relatrice, a meno che io non abbia davanti

Senatrice Simeoni, ha un testo che possa essere considerato un ordine del giorno, secondo le osservazioni?

proponente, presentato adesso, dice: impegna - «a valutare l'opportunità di», questa è la mia proposta - a intraprendere tutti gli opportuni provvedimenti affinché i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta siano tenuti a fornire ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori tutte le informazioni necessarie al fine di comprendere le peculiarità cliniche ed epidemiologiche delle pratiche vaccinali di cui al comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, prevedendo altresì che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori debbano sottoscrivere un apposito modulo predisposto dal Ministero della salute entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge di cui dichiarato di aver ricevuto l'informativa in merito alle pratiche vaccinali di cui al comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame. Naturalmente l'impegno al Governo prevede una riformulazione con la formula "a valutare l'opportunità di".

Per la verità, sto intervenendo per comprendere un fatto. C'è tutto un effluvio di emendamenti e di ordini del giorno per stabilire chi debba spiegare ai genitori

i dati dell'Aifa, che è l'ente preposto a valutare e a rendere note le complicanze gravi e meno gravi, non sono stati citati né dalla relazione, né dal relatore, né dalla signora Ministro. Adesso c'è tutta la storia su chi debba raccontare ai genitori le complicanze, quando qua noi stiamo procedendo alla cieca, cioè con la pervicace volontà di non rendere edotta l'Aula...

«sul proprio sito, sulle nuove vaccinazioni effettuate, sui progressi nella copertura vaccinale della popolazione, sulle modalità di approvvigionamento dei vaccini e sui loro costi». Sono dati che normalmente il Ministero mette sul sito, non c'è alcuna spesa.

Il comma 7 prevede che l'Assemblea possa deliberare, su proposta di otto senatori «in relazione a situazioni sopravvenute ed urgenti,

ci sono state ripetute occupazioni di filiali della Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca da parte dei cittadini truffati dalle precedenti amministrazioni bancarie. Vi sono stati dei tentativi di suicidio,

essa propone di introdurre nuove norme volte a erogare sanzioni adeguate riferibili all'esercizio dell'azione di responsabilità,

In secondo luogo, la mozione si propone di ampliare la platea degli obbligazionisti beneficiari del previsto fondo di solidarietà.

fiducia e, sostanzialmente, non ci sarà la possibilità di avviare alcuna discussione parlamentare sulle modifiche necessarie a tale decreto-legge.

Non si deve sapere che il decreto-legge, di fatto, nega giustizia ai risparmiatori, truffati e traditi dagli amministratori di queste due banche. Non si deve sapere che il decreto-legge non fa nulla per far pagare chi ha sbagliato

Signor Presidente, il nostro Gruppo è stato quello che per primo ha presentato una mozione su questa materia, che è stata sottoscritta, tra l'altro, da

per considerare l'importanza di questo argomento, che va al di là della materia che tratta, ed è la seguente: in realtà le mozioni riprendono il contenuto di un emendamento concordato da tutti i Gruppi nella Commissione bilancio della Camera dei deputati. Tale emendamento non è stato poi messo ai voti, perché in quel ramo del Parlamento è intervenuto un voto di fiducia.

Tutto questo mi porta a dire, signor Presidente, che l'intervento che mi ha preceduto è sicuramente fondato nelle sue argomentazioni e anche nelle sue richieste. La delicatezza della materia, che d'altra parte è stata illustrata, mi porterebbe a suggerire, anche a chi mi ha preceduto, una inversione delle richieste. Secondo me, la principale richiesta dovrebbe essere un impegno

la possibilità di ricomprendere quell'emendamento, che è stato cassato, e per stabilire un tempo perché la Camera possa nuovamente tornare a occuparsi della materia. Ma ripeto, signor Presidente, questo sta alla sensibilità

durante la seduta. Si tratta di argomenti di estrema delicatezza e, tra l'altro, io li considero anche in relazione a quelli che sono stati i lavori svoltisi oggi pomeriggio in Commissione finanze. Quindi, esse

decisione e qualsiasi opinione non potrà avvenire che dopo aver esaminato i documenti. Debbo dire, in modo molto superficiale, che io non vedo cosa c'entri la Conferenza dei Capigruppo. Qui noi abbiamo delle mozioni su cui dobbiamo esprimerci. Poi, avremo un provvedimento di

a nome del Gruppo Lega Nord per esprimere il nostro voto favorevole alla calendarizzazione e alla discussione immediata delle mozioni relative alla alla questione, molto spinosa della responsabilità di chi ha condotto banche ormai in crisi quasi

perché in quel provvedimento si evidenzia ancora, da parte del Governo, la volontà di colpire i risparmiatori, di non assicurare adeguati indennizzi,

che fanno ricadere esclusivamente sui risparmiatori responsabilità che non sono loro ma di altri, è un atteggiamento inaccettabile, che condanniamo, e che ha visto protagonisti prima il Governo Renzi e ora il Governo Gentiloni Bisognava invece prendere atto del fatto che, a fronte di una crisi sistemica dell'Italia con un calo del prodotto interno lordo del 10 per cento, la crisi bancaria è esclusivamente una conseguenza di politiche sbagliate da parte dei Governi che si sono succeduti negli ultimi sei

Non si possono penalizzare esclusivamente quei cittadini che hanno riposto la propria fiducia in istituti bancari che sono stati gestiti male e che si sono trovati in seria difficoltà a causa di questa crisi epocale e non passeggera che riguarda l'intero Paese, la sua economia e solo di conseguenza il sistema bancario. Ci sono crediti inesigibili non necessariamente perché

nella difficoltà di farle sopravvivere, non hanno avuto alcuno scrupolo nel sottoporre a ignari risparmiatori prodotti che non dovevano essere loro proposti e incentivati.

mozioni è delicata e importante, perché richiede all'Assemblea di intervenire in una discussione che in qualche modo impatta e interferisce sull'esame del decreto-legge n. 99 del 2017. D'altra parte, anche se questa procedura è anomala, ha una sua motivazione nel fatto che noi abbiamo la consapevolezza che quel provvedimento arriva praticamente con un'impossibilità di modifica, quindi il Senato non ha, di fatto, altra possibilità di esprimersi

Siamo di fronte a mozioni che in larga parte riprendono proprio il contenuto di un emendamento che il mio Gruppo, e in particolare i colleghi Zoggia, Bersani e Ragosta hanno presentato alla Camera, che poi è stato condiviso anche dagli altri Gruppi ma di cui ovviamente io rivendico la paternità. Questo emendamento non è poi stato fatto proprio, diversamente da quanto si pensava, dal relatore, quindi di fatto non è stato votato.

seguano l'interdizione dai pubblici uffici, l'impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione, l'impossibilità di mettersi alla guida di un'altra banca. Si tratta di un punto assolutamente cruciale, perché chi svolge la funzione di amministratore di una banca svolge una funzione di pubblico

Devo segnalare anche che oggi, in audizione in Commissione finanze, ho chiesto al ministro dell'economia Padoan cosa pensasse di questo tema ed il Ministro ha risposto che sarebbe assolutamente d'accordo con una norma che prevedesse quello che anche noi suggerivamo e, forte anche di questo generico sostegno, credo sia opportuna una discussione del tema in quest'Assemblea, anche nella forma immediata che è stata richiesta, ovviamente secondo modalità che permettano a tutti i colleghi di poter approfondire i contenuti delle proposte e di arrivare quindi ad un voto consapevole.

ove i commissari liquidatori esercitassero l'azione di responsabilità, il giudice, qualora accogliesse la domanda, condannasse sempre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Per la rilevanza e per lo spirito di questo emendamento, riteniamo sia assolutamente necessario discutere queste mozioni in modo tale da impegnare il Governo a recuperare

accolla tutti i costi delle operazioni di salvataggio alla collettività e regala invece le due banche, ripulite dalle sofferenze,

Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà a favore della calendarizzazione di questa mozione, che naturalmente potrà essere affiancata da altre mozioni. Noi probabilmente ne presenteremo una per conto nostro, perché riteniamo importante che ci sia il perseguimento delle responsabilità

un messaggio rivolto a coloro che oggi amministrano delle banche. Noi riteniamo giusto che vengano salvati i risparmiatori, nella misura in cui hanno investito in titoli sicuri o presentati come tali (a maggior ragione se hanno semplicemente dei depositi), ma riteniamo altresì che ci debba essere una responsabilità da parte di chi, con il proprio comportamento (dipende anche

quotidianità, con le misure che vengono fatte passare come indispensabili e urgenti (mentre qui parliamo di miliardi), è importante che ci sia un approfondimento delle responsabilità Naturalmente chi non ha responsabilità e si è comportato bene non può essere punito per il solo fatto di aver fatto parte dell'amministrazione di una banca che poi ha avuto dei risultati fortemente negativi.

i prestiti e si garantiscono le linee di credito, è assai probabile che diventino sofferenze; pertanto è evidente che lì c'è una responsabilità. siamo pertanto a favore di questa mozione, che assieme ad altre deve sottolineare questo aspetto. È giusto salvare i risparmiatori, a tutela non soltanto degli stessi, ma per la tenuta in generale del sistema bancario del nostro Paese, che è fatto di di diversi elementi, due dei quali sono una buona amministrazione e la consapevolezza che chi si comporta male poi verrà punito. Altrimenti sarebbe come un incentivo ad altri amministratori di banche a comportarsi nello stesso modo, avendone molto probabilmente qualche vantaggio personale. Infatti, quando si presta qualche decina di milioni di euro a persone cui non si dovevano prestare i soldi, è abbastanza verosimile che da parte di queste persone ci sia una riconoscenza indebita, magari molto nascosta. prevenire e dunque perseguire coloro che si comportano male, a tutela dei contribuenti e a tutela del sistema bancario italiano. Signor Presidente, il voto che ci accingiamo a esprimere è volto a inserire all'ordine del giorno la discussione delle mozioni. Avrei preferito, per una ragione di stile, che ci fosse un impegno unanime unanime dell'Assemblea ad assolvere a questo compito all'interno di una Conferenza dei Capigruppo; avremmo potuto così armonizzare questa discussione rispetto al decreto-legge sulle banche. È assolutamente evidente che, rispetto all'armonizzazione, tra maggioranza e opposizione vi siano dei

Colgo l'occasione per annunziare che in Commissione finanze noi reitereremo la richiesta di audizione dell'amministratore delegato di Unicredit Ghizzoni

la tutela del risparmio, il credito alle imprese e alle famiglie, il sistema bancario e il centro della vita economica di un sistema complesso come quello di una grande democrazia economica quale è quella italiana.

di difficile accesso per la varietà delle argomentazioni usate per illustrarle e per la complessità del dispositivo, possano essere messi in discussione nell'Aula del Senato con l'urgenza che è stata richiesta. Penso che si tratti di argomenti che debbano essere ben soppesati, che richiedano una grande prudenza nei modi e nei tempi con cui vengono maneggiati e che sia, quindi, non prudente - uso un'espressione

È stata messa in evidenza la connessione temporale, che, d'altra parte, è sotto gli occhi di noi tutti, tra il contenuto di queste mozioni e quello di un decreto-legge che verrà all'esame

che versa tutt'ora in gravi difficoltà; difficoltà che hanno molto allarmato l'intera economia italiana, a cui è stato posto rimedio da parte del Governo con un decreto-legge che è stato - possiamo dire - coordinato con il lavoro della Commissione europea nei minimi particolari.

Se non ho mal compreso, il senatore Quagliariello ha sostenuto la tesi che la calendarizzazione della discussione di queste mozioni debba essere decisa dalla Conferenza dei Capigruppo. Credo che questa sia un'indicazione seria. Quando la Presidenza del Senato riterrà opportuno e necessario che la Conferenza dei Capigruppo venga convocata, questo è un argomento classico,

Personalmente ho molto apprezzato la posizione che, in tema di responsabilità degli amministratori delle banche, oggi abbiamo ascoltato da parte del ministro Padoan in Commissione finanze proprio qui al Senato.

Chiedo all'Assemblea di considerare con attenzione la proposta del senatore Quagliariello perché l'importanza e la delicatezza dell'argomento francamente credo che sconsiglino l'immediata discussione di un

Signor Presidente, apprezzate anche le considerazioni del senatore Zanda, io credo che sia più opportuno votare sulla calendarizzazione di queste mozioni queste mozioni che non hanno alcun contenuto relativo alla situazione economica del nostro Paese. Non so se il presidente Zanda le abbia lette. Si tratta di decidere se i responsabili di crimini gravissimi devono andare in galera e se devono subire delle sanzioni

vota per alzata di mano?

alla soglia dei cento anni, e la sua lunga, intensa e operosa vita, fatta di impegno politico costante e di attiva presenza sulla scena politica...

ricordare la sua lunga, intensa e operosa vita, fatta di impegno politico costante e di attiva presenza sulla scena politica italiana e nella quotidianità della sua città. La sua esistenza e la sua cultura politica sono state un tutt'uno con la storia del socialismo italiano, del quale è stato sicuramente un influente militante e un animatore instancabile. Alle esequie hanno ricordato la sua carriera politica il sindaco di Viareggio e l'amico Valdo Spini; e non basterebbero ore per raccontare della sua operosa attività nazionale e dell'influenza che ha sempre avuto nella sua Versilia e nella sua città. Ma lo voglio ricordare, in particolare, per un fatto che forse più di altri rappresenta la sua personalità e la sua attività. Fu il primo, tra i Ministri del Governo in carica nell'anno della drammatica alluvione di Firenze, quel 4 novembre, a raggiungere la città. La raggiunse grazie a un mezzo anfibio dell'Esercito e si insediò in prefettura. Come Ministro fu lui ad adottare i provvedimenti che permisero alle aziende fiorentine e alla città di rinascere. Politica, arte e cultura sono stati sempre i tre cardini intorno ai quali ha speso una lunga vita, intensa, battagliera, generosa e attiva fino ai suoi ultimi giorni, alla soglia dei cento anni. Permettetemi, dunque, di ricordare gli aspetti che ho conosciuto di lui, in una delle fasi in cui, più che novantenne, non aveva perso niente della combattività che aveva caratterizzato tutta la sua vita. Aveva sempre pronto nel cassetto un "libro dei sogni", fatto però di progetti concreti, e non si dava pace se non riusciva a farli mettere in cantiere. Da quando aveva concluso la sua attività istituzionale si era dedicato soprattutto alla cultura e all'arte, continuando a coltivare intensamente i rapporti con artisti, musicisti, intellettuali, con l'istituto Sant'Anna di Pisa e con la Fondazione Turati, con l'ambizione di contribuire a sprovincializzare la cultura italiana, a partire dalla sua città. Ha infatti rivolto tanta parte del suo impegno a superare ogni forma di campanilismo della della cultura italiana e versiliese auspicando quella visione più ampia e unitaria che ancora oggi fa tanta fatica a radicarsi. La nostra città gli deve molto, non solo per la donazione della vasta collezione di arte contemporanea, che si era costruito negli anni, ma anche per l'impegno dedicato alla Galleria d'arte moderna e contemporanea cui ha profuso tante energie e dove è riuscito a realizzare il centro internazionale della grafica. Durante i nostri incontri, nei quali non ci scordavamo di litigare perché le sue idee faticavano a essere accolte con entusiasmo dalla classe dirigente viareggina del momento, finiva sempre per farsi portare dalla signora Vera, la moglie, l'ultimo studio, l'ultimo progetto che non riguardava solo la cultura, ma anche il turismo, come la sua profonda convinzione della necessità di destagionalizzare con grandi eventi da accompagnare al carnevale, come il Festival del mare e il Festival d'inverno. Come si faceva a non dargli ragione, a non inchinarsi di fronte a tanta lucidità, nonostante gli anni, a tanta voglia di progettare il futuro della sua città e di guardare avanti? Da questi incontri si usciva estenuati, ma sicuramente arricchiti e spronati a combattere per veder tornare a risplendere quella quella Viareggio che tanto amava. Dunque, non posso che salutare dicendo: grazie Giovanni per tutto quello che hai fatto e soprattutto per quello che hai sognato per la nostra città, ti assicuro che ce la stiamo mettendo tutta per veder realizzati tanti di quei progetti che, in fondo, non erano sogni, ma cose concrete che tutti coloro che amano Viareggio e la Versilia condividono, i quali hanno però bisogno di quella generosa battagliera volontà di quella determinazione che hanno caratterizzato tutta la tua vita. Grazie ancora, ci mancherai.

Ringrazio la Presidenza per il pronto intervento, anche a seguito di quello che poi è avvenuto nei giorni seguenti. I Ministri si sono mossi

nelle ore a maggior rischio, ossia quelle notturne, quando le operazioni di protezione civile sono sospese. Voglio ricordare che ultimamente - ahimè

vogliamo capire bene cosa sta accadendo in Italia, perché non credo a quello che normalmente viene detto quando ci sono questi incendi e si chiama

Come preannunciato nel mio precedente intervento, torno a denunciare il fatto che sono ancora rimaste inevase le interrogazioni del Gruppo della Lega Nord

statistico giornaliero è scomparso il numero dei richiedenti asilo/ rifugiati presenti nel sistema di accoglienza, nei centri di prima accoglienza, nei centri di accoglienza straordinaria, negli *hotspot* e nei posti del Presidente, l'accoglienza fa la parte del leone nel costo complessivo che lo Stato italiano sostiene: si tratta di 4,7 miliardi di euro, come ha detto il cento afferisce al sistema di accoglienza. L'assenza di tali numeri, relativi alle presenze nel sistema di accoglienza, insospettisce noi della Lega Nord e la riteniamo una grave mancanza di trasparenza ripeto - non tanto nei confronti del nostro Gruppo, ma nei confronti dei cittadini italiani. Gli ultimi dati disaggregati, che come Lega Nord siamo riusciti ad ottenere e che risalgono a maggio 2015, ci parlano di circa 182.000-183.000 presenze secondo i nostri calcoli, mancano almeno 50.000-60.000 presenze. Secondo noi dovremmo registrare nel sistema di accoglienza circa 240.000 presenze, che sono un numero importante. Sottolineo che i ricollocamenti

la gran parte dei clandestini, per un tempo medio di due anni, e buttiamo fuori quei pochi profughi che vengono nel nostro Paese. Questo, signor Presidente, è un paradosso su cui il Ministero dell'interno deve fare chiarezza, anche se riteniamo che le motivazioni di questa forte discrepanza tra i numeri non siano solo legate a coloro che, ottenuto lo *status*, vengono immediatamente sbattuti fuori, ma ci sia qualcosa d'altro.